finestra"). Comunico che, in data 15 febbraio 2023, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di senatori Segretari. Ai sensi della disposizione transitoria del Regolamento del Senato per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura, i Gruppi Azione-Italia Campobase, Sud Chiama Nord) hanno avanzato la richiesta di procedere all'elezione di due ulteriori senatori Segretari. Su tale richiesta si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Presidenza per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulta alterato il rapporto numerico in seno al Consiglio di Presidenza tra i componenti dei Gruppi di maggioranza e dei Gruppi di opposizione. Si procede pertanto, ai sensi dell'articolo 3 della citata disposizione transitoria, alla contemporanea elezione di un ulteriore senatore Segretario appartenente ai Gruppi di maggioranza. Ai sensi del comma 4 della medesima disposizione transitoria, ciascun senatore può scrivere sulla scheda un

per i Gruppi di maggioranza, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento, a parità di voti è eletto il più anziano di età. Dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte, come vedete, due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna, all'uscita della cabina stessa.

De Carlo, De Cristofaro,

Fina, Floridia Aurora,

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, le dichiarazioni rese da Nina Corradini e da altre ex atlete della nazionale di ginnastica ritmica sulle pressioni psicologiche subite, anche attraverso un controllo ossessivo del loro peso, hanno portato alla luce uno scenario preoccupante, che non è stato ignorato. Il rischio di far nascere disturbi psicologici e alimentari, che mettano a repentaglio lo stato di salute fisico e mentale degli atleti e allontanino i giovani dello sport, è intollerabile. Ho dichiarato in modo inequivocabile, nei giorni successivi, che nessuna medaglia, per quanto fattore di orgoglio nazionale o soddisfazione personale, potrà mai giustificare trattamenti degradanti e lesivi del benessere psicofisico degli atleti e delle atlete, specialmente se minorenni, al solo scopo di ottenere da loro migliori prestazioni. Nel rispetto dei ruoli, spetterà alle autorità competenti, non solo sportive, effettuare gli opportuni accertamenti, appurare le dimensioni effettive della vicenda e le relative responsabilità e comminare le conseguenti sanzioni.

e del *safeguarding officer*, organismo promosso dalla federazione proprio per favorire la raccolta di eventuali segnalazioni di comportamenti impropri. A questo proposito, ho registrato un'immediata attivazione delle due strutture federali, ma posso anche segnalare il nostro impegno per rafforzare e promuovere al meglio le misure che abbiamo già adottato, a tutela e garanzia della salute psicofisica delle nostre atlete e dei nostri atleti di tutte le discipline e, se necessario, adottarne altre, tenendo conto, senatrice Valente, anche delle sue e delle vostre proposte, per le quali vi ringrazio, a partire dalla creazione di un centro di ascolto terzo, da noi promosso e coordinato, con un numero verde dedicato. Credo che in ogni caso sia opportuno informarvi che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha già istituito un tavolo tecnico con 26 enti e associazioni, per la costituzione e la promozione di una struttura finalizzata a rafforzare la tutela dei minori nel mondo dello sport, con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi e l'obiettivo di garantire a tutti i giovani atleti e atlete di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro. Per favorire la diffusione di questa iniziativa, frutto della collaborazione tra chi ha la responsabilità di normare e chi ha la responsabilità di formare e seguire i giovani nelle realtà locali, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione, il cui *slogan* è «Battiamo il silenzio». È stata inoltre predisposta una piattaforma *web* contenente documenti e informazioni facilmente accessibili e utili strumenti di formazione fruibili in qualsiasi momento da parte del personale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché dei docenti ed educatori, oltre all'indicazione delle istituzioni alle quali potersi rivolgere e dei numeri utili per eventuali segnalazioni. Il nostro Dipartimento per lo sport ha inoltre supportato il progetto di ricerca sugli abusi nel contesto sportivo che l'organizzazione di volontariato «Il cavallo rosa/ Change the game» ha commissionato alla di ricerca Nielsen per individuare la dimensione realistica del fenomeno, anche la luce delle recenti denunce. A tal fine è stato scelto un campione di 1.400 individui di età compresa tra i diciotto e i trent'anni che prima dei diciotto abbiano praticato attività sportive individuali o di gruppo con un'associazione sportiva; sono state realizzate venti interviste. Da ciò è nato il progetto sulla cultura dell'atleta e il sondaggio sul clima, con l'obiettivo d'indagare sulle dinamiche alla base della violenza interpersonale contro i minori all'interno della pratica sportiva, informare l'opinione pubblica sull'entità del fenomeno e sui disagi da essa provocati, sensibilizzare quanti lavorano nell'ambito dello sport organizzato e fornire un supporto alla creazione di politiche volte a prevenire il fenomeno della violenza nella pratica sportiva, nonché ad accrescere il *corpus* di indagini legate a tale fenomeno. Devo anche segnalare che il tema delle molestie nel mondo dello sport è stato al centro dell'incontro realizzato due mesi fa con la Presidente dell'Associazione nazionale atlete, che ha proposto insieme ad altre cinque organizzazioni *partner* il progetto europeo «Fair coaching», con l'obiettivo di fornire conoscenza e strumenti utili agli allenatori e alle allenatrici al fine di prevenire e contrastare comportamenti sessisti, violenti e discriminatori e garantire un ambiente sportivo sano e stimolante. Anche grazie a questo progetto non faremo mancare il nostro sostegno. Con la medesima finalità, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, assieme all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e alla Scuola dello sport - sport e salute ha messo a disposizione dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive un *vademecum,* al fine di accompagnarli e supportarli nelle loro attività a sostegno del percorso di crescita dei minori impegnati nelle attività sportive e rendere uniforme la capacità di risposta del mondo dello sport su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal diverso contesto organizzativo. I tecnici e i dirigenti sportivi rappresentano un fondamentale punto di riferimento non soltanto per l'acquisizione di competenze, ma anche per il trasferimento di valori educativi e di uno stile di vita sano, nonché per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, affinché le atlete e gli atleti possano godere appieno del loro diritto. Considero quest'occasione anche una preziosa opportunità per rappresentare e rilanciare il nostro impegno comune per consolidare la centralità del valore del rispetto in tutte le sue declinazioni, a partire dai comportamenti e dal linguaggio nello sport e non solo. Di fronte a questo rinnovato impegno, sarà fondamentale una diffusa e convinta collaborazione che per primo non posso che riconfermare di fronte a voi.

Ci teniamo a sottolineare che il tema della violenza contro le donne è un tema generale, del quale anche quest'Assemblea e questo Parlamento si occupano a 360 gradi; tuttavia, il fatto che si consumino episodi di violenza in un mondo come quello dello sport, che dovrebbe lavorare per garantire un maggiore benessere psicofisico soprattutto di tanti ragazzi e di tante ragazze, è qualcosa che preoccupa e che deve richiamare l'attenzione di tutti quanti noi. È un impegno che dovrebbe vederci impegnati

Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Martella segnala la sosta, protratta per giorni nelle adiacenze della questura di Treviso, di diversi richiedenti asilo in attesa di essere inseriti nel circuito dell'accoglienza, chiedendo iniziative al fine d'individuare una soluzione per ospitarli in maniera dignitosa e velocizzare le procedure per il riconoscimento del diritto di asilo. La prefettura di Treviso, interessata sulla vicenda, ha comunicato che la problematica segnalata nell'interrogazione è stata già risolta. Infatti, tutte le persone che sostavano davanti alla questura sono state accolte nei centri di accoglienza straordinaria, i CAS, presenti nella provincia. In particolare, si trattava di 30 richiedenti asilo provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh, giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, che sono stati ospitati nelle strutture di accoglienza tra il 22 dicembre 2022 e il 9 gennaio scorso. Su un piano più generale, la prefettura ha evidenziato che, dal gennaio 2022 all'inizio del gennaio 2023, sono stati raccolti nei centri di accoglienza straordinari della provincia 109 migranti, per lo più di origine pakistana, presentatisi spontaneamente presso la locale questura per avanzare richiesta di protezione internazionale. Al riguardo, va rilevato che i tempi d'attesa per gli inserimenti nel circuito dell'accoglienza si sono prolungati a causa dell'afflusso dei migranti e, in particolare, dei consistenti arrivi autonomi dalla rotta balcanica, che come tali non sono preventivabili in anticipo e che, pertanto, hanno determinato la progressiva saturazione dei posti disponibili nelle strutture del sistema di accoglienza provinciale. In tale contesto, la prefettura di Treviso si è sempre prontamente attivata per eliminare ogni criticità e mitigare situazioni di disagio al fine di assicurare, in particolare, l'immediata accoglienza delle persone più vulnerabili. La prefettura ha inoltre rappresentato che, alla data del 13 gennaio 2023, nella Provincia di Treviso sono attivi otto centri d'accoglienza straordinaria nei quali sono ospitate 972 persone, con un incremento di 380 unità rispetto alle 502 presenze registratesi al 1° gennaio dello scorso anno. Si segnala inoltre che, nel corso del 2022, le richieste di protezione internazionale sono state 692, a cui si sono sommate le pratiche di rinnovo dei titoli di soggiorno in attesa della decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e quelle in attesa della pronuncia del tribunale di Venezia in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego dei medesimi titoli. Per quanto riguarda infine la tempistica dell'*iter* per il riconoscimento del diritto d'asilo, la locale sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha assicurato che le relative procedure si svolgono nel pieno rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Signor Presidente, voglio ringraziare il sottosegretario Molteni per la risposta, di cui prendo atto. In effetti, il caso è stato risolto nel corso delle settimane precedenti, ma è del tutto ovvio che, quando ho presentato quest'interrogazione, la stampa nazionale e locale aveva posto in grande risalto la condizione di questi migranti che, in attesa della definizione della loro pratica di richiedenti asilo, vivevano e dormivano davanti alla questura di Treviso. Penso che

nel trovare soluzioni, la verità è che non si esercita la responsabilità pubblica che bisogna esercitare. Purtroppo, come lei stesso ha ricordato, i tempi per l'evasione delle pratiche dei richiedenti asilo sono molto lunghi: più o meno dodici mesi, più altri sei per la concessione del permesso di soggiorno. È per questo che riteniamo che servano più personale presso le questure e le prefetture per poter espletare queste pratiche

in Veneto e non solo. La nostra richiesta era proprio indirizzata su questo doppio versante: aumentare, da un lato, il personale; dall'altro, dall'altro, la disponibilità dei posti, perché queste persone non si trovino a vivere in situazioni di degrado. Mi auguro che le risposte che sono venute e le rassicurazioni da parte della prefettura e della questura di Treviso vadano in questo senso e che soprattutto si possano diminuire fortemente i tempi d'attesa.

i senatori interroganti chiedono al Ministro della cultura quali iniziative intenda intraprendere al fine di sopperire alla carenza di personale del museo archeologico di Muro Lucano, in provincia di Potenza, e scongiurarne la chiusura. Al riguardo occorre evidenziare come il Ministro della cultura abbia tempestivamente informato i propri uffici del problema della carenza di personale presso il museo lucano, recependo le istanze già rappresentate dal sindaco della città di Muro Lucano, Giovanni Setaro, preoccupato della sorte del museo archeologico che, nonostante l'esiguità dei visitatori giornalieri, costituisce comunque il centro di riferimento per la conoscenza della storia antica del territorio del Marmo-Platano-Melandro. Per la verità, le difficoltà di gestione del museo archeologico nazionale di Muro Lucano non sono purtroppo isolate, essendo invece condivise da altri istituti museali statali, inclusi quelli della Regione Basilicata. Al fine di far fronte a tali criticità e garantire la funzionalità degli istituti culturali, il Governo ha presentato di recente un emendamento al decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, cosiddetto proroga termini, attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge,

per il reclutamento di complessive 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella seconda area posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

Come noto, il disegno di legge dovrà essere approvato entro il prossimo 27 febbraio: una volta concluso l'*iter* di conversione, lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso innanzi citato potrà fornire nuove risorse di personale a enti e istituti di cultura, incluso il museo di Muro Lucano, aiutando a sopperire alle attuali carenze. ringrazio il Governo e il sottosegretario Mazzi per la risposta, anche al nome del collega Rosa, quale primo firmatario dell'interrogazione.

di cui abbiamo parlato oggi, questo sia l'inizio di una procedura che cerca di sanare una carenza di organico che, come dicevo prima, non si esaurirà neanche con l'ingresso

il 25 gennaio sono intervenuta in quest'Aula per chiedere al Ministro della cultura di tutelare il museo archeologico nazionale di Muro Lucano, che rischiava di chiudere a causa dell'esiguità del personale in servizio, a cui si sarebbe aggiunta la quiescenza prossima di alcuni lavoratori. È una richiesta che ho inteso rafforzare depositando un'interrogazione parlamentare e sollevando il caso sulla stampa nazionale. Assieme ai sindaci di Muro Lucano e dell'area interna Marmo Platano abbiamo cercato in tutti i modi di preservare un'eccellenza della nostra terra, ritenendo che alcuni beni, diritti e servizi essenziali non debbano avere colore politico. Pertanto, mi ritengo soddisfatta della risposta fornita: sapere che il Ministero della cultura abbia accolto la richiesta di salvare il sito culturale, individuando le unità di personale necessarie - come ci ha riportato,

e quanti usufruiscono del meraviglioso complesso museale. Attenzione: colgo l'occasione per evidenziare che la soddisfazione è solo sul caso specifico, e cioè sul museo di Muro Lucano. Nel complesso, infatti, i siti culturali del Paese e in particolare delle aree fragili del Mezzogiorno

sottosegretario Mazzi, con riferimento all'interrogazione parlamentare 4-00160, depositata in data 24 gennaio 2023, avente ad oggetto le istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato. Sul punto ricordo che, alla luce degli attuali criteri stabiliti dal Ministero, il 40 per cento degli stanziamenti è stato ripartito tra gli istituti del Settentrione, il 51 per cento tre gli istituti del Centro Italia e appena il 9 per cento tra quelli del Mezzogiorno. E proprio la Basilicata, Regione di cui stiamo discorrendo, per il triennio 2021-2023 non ha ottenuto nemmeno un euro, mentre altre, come la Toscana o l'Emilia Romagna, terra nativa dell'ex ministro della cultura Franceschini, hanno ottenuto finanziamenti rispettivamente per 33 e 20 siti culturali. Attendo dunque di sapere se sarà possibile ristorare le Regioni che non hanno ottenuto finanziamenti, come appunto la Lucania, e se il Ministero intenderà modificare i requisiti di accesso al finanziamento, cercando soprattutto di eliminare gli eventuali vincoli che hanno impedito ad alcune Regioni di presentare domanda. Questo è importante: i requisiti e i parametri sono da cambiare. In attesa di una risposta, ringrazio per l'attenzione

finestra") sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari a fissione sul territorio italiano.

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, si rappresenta quanto segue: ai fini del raggiungimento di una sempre maggior sicurezza e autonomia energetica, nonché in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica previsti a livello europeo, è necessario operare in direzione della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ovvero soluzioni volte a soddisfare le esigenze del Paese in modo coerente e sufficiente. Pertanto, occorre dare una risposta concreta sia alle crescenti domande di energia, sia alla necessità di ridurre le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi del *green deal* e con l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente. La crisi energetica, acuitasi con il conflitto russo-ucraino, ha posto in evidenza, non solo a livello nazionale, la necessità del raggiungimento dell'indipendenza energetica, riportando all'attenzione del dibattito pubblico anche il tema dell'energia nucleare, considerato che allo stato attuale le fonti rinnovabili devono ancora esprimere tutto il loro potenziale attraverso l'implementazione diffusa degli impianti, dei sistemi e delle modalità di produzione e consumo, al fine di poter sopperire autonomamente e pienamente al fabbisogno energetico. Premesso quanto sopra, si rammenta che una prima rinuncia nel territorio nazionale all'utilizzo dell'energia nucleare da fissione per la produzione di energia elettrica è avvenuta in conseguenza del primo *referendum* abrogativo del 1987, che ha portato all'arresto sia delle centrali nucleari ancora attive sia degli impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché all'interruzione dei lavori di costruzione delle centrali di Montalto di Castro e di Trino 2, entrambe peraltro mai entrate in funzione. Successivamente, il tentativo più recente da parte del Governo di rilanciare la produzione elettronucleare è avvenuto mediante il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante misure per la disciplina della localizzazione, realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Come noto, l'esito del *referendum* del giugno 2011 ha tuttavia sancito nuovamente l'abbandono dello sviluppo nucleare in Italia per la produzione di energia elettrica, con la conseguente abrogazione del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per la parte relativa alle procedure realizzative di nuovi impianti di produzione di energia elettrica nucleare e fabbricazione di combustibile nucleare. Pertanto ad oggi l'utilizzo di reazioni di fissione nucleare per la produzione di energia elettrica (e conseguentemente la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di reattori nucleari) non è previsto dalla normativa. Inoltre, in ragione dell'abrogazione della parte del decreto legislativo n. 31 del 2010 relativa alla produzione di energia tramite fonte nucleare, ad oggi non esiste un impianto regolatorio nazionale per l'autorizzazione di qualunque delle fasi citate. Pur tuttavia, la ricerca sul nucleare di quarta generazione, sugli *small modular reactor* (SMR) e sulla fusione nucleare è molto attiva a livello mondiale, poiché è considerata potenzialmente in grado di apportare significative soluzioni alle questioni legate alla generazione sostenibile di energia. Diversi studi e pratiche di ricerca applicata sugli impatti ambientali e sugli effetti sulla salute sono ampiamente considerati, così come la sicurezza e la sostenibilità. L'Italia, tramite i suoi istituti di ricerca, le università e alcune società private, è impegnata da tempo nella ricerca sul nucleare di quarta generazione, sui piccoli reattori modulari e sui reattori modulari avanzati. Nell'ambito dei progetti in fase di studio, si evidenziano programmi quale il NuScale, ovvero un SMR il cui concetto di generatore di vapore è testato presso Siet (società partecipata da Enea), e ancora il Rolls-Royce SMR, che ha in essere interlocuzioni con Siet, Enea e Ansaldo nucleare per la valutazione sperimentale in Italia.

supportato dal consiglio internazionale Falcon, del quale attualmente sono membri Ansaldo nucleare ed Enea per l'Italia, il centro di ricerca Rez per la Repubblica Ceca e l'Istituto per la ricerca nucleare per la Romania. La stessa Enea partecipa insieme ad Ansaldo nucleare nel supporto alla realizzazione di diversi impianti sperimentali nell'ambito del programma AMR-UK. Per quanto concerne invece il reattore modulare avanzato e sviluppato dalla *start-up* Newcleo, si specifica che quest'ultimo si basa su tecnologia Enea e viene sviluppato presso le infrastrutture dell'ente stesso, anche grazie a investimenti che ammontano a oltre 50 milioni di euro. Ad ogni buon fine, si ritiene necessario guardare con attenzione e senza pregiudizi a tutte le soluzioni in grado di favorire il processo di decarbonizzazione e d'indipendenza energetica, attraverso un approccio improntato alla neutralità tecnologica. In particolare, nell'ambito della fissione nucleare, è in corso uno sforzo a livello mondiale per lo sviluppo in tempi rapidi (entro il decennio) di diversi tipi di SMR, piccoli reattori modulari già autorizzati o in fase di autorizzazione da parte di alcuni Paesi, adatti per vari utilizzi (energetici, teleriscaldamento, produzione di energia e calore in zone di difficile accesso, generazione di idrogeno, eccetera). In relazione ai tempi di costruzione di impianti nucleari a livello internazionale, si stimano intorno ai quattro-sei anni per gli SMR e tra otto e dieci anni per i reattori di grande potenza. Per quanto riguarda valutazioni più precise sui tempi di costruzione, nonché sui costi, inclusi quelli relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti, si specifica che dipendono principalmente dalla tipologia di reattori utilizzati, atteso che gli studi attuali si basano pressoché esclusivamente sul nucleare esistente, quasi esclusivamente di seconda generazione, e comunque tengono in considerazione l'intero ciclo nucleare, incluso lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Infine, nel rappresentare come le energie rinnovabili variabili presentino tuttora il problema di non coprire a sufficienza il carico di base di generazione in quanto intermittenti per loro natura, non va assolutamente sottovalutato l'impegno profuso dalle primarie istituzioni di ricerca pubbliche e private, nonché dai principali operatori economici, nel sostenere la ricerca nazionale verso soluzioni tecnologiche innovative per la massimizzazione dello sfruttamento delle suddette fonti e dei sistemi di accumulo. A tale ultimo proposito, si sottolinea come il volume di risorse allocate attraverso il PNRR, il Piano triennale della ricerca e di sistema elettrico e l'iniziativa multilaterale Mission Innovation risulti particolarmente significativo, coinvolgendo le principali istituzioni di ricerca nazionali nella conduzione di attività innovative volte alla sempre maggior valorizzazione delle energie rinnovabili e nell'adozione di tecniche efficienti e affidabili che possano altresì valorizzare le filiere nazionali.

Perché non è che lei non abbia voluto dire al Parlamento e al Paese dove volete realizzare la o le centrali nucleari di cui si è parlato in campagna elettorale, con quali tempi e con quali costi. Lei correttamente ha detto che non c'è niente.

Effettivamente, si tratta di una libera discussione buona per i laboratori di ricerca avanzata, così come indistintamente per i bar sport. Voi invece siete costretti in un ruolo su cui le consiglio una riflessione, anche di carattere etimologico. Ministro deriva da *minus*, quindi è un ruolo umile. Siete chiamati ad amministrare umilmente la cosa pubblica, concretamente. La ricerca, che lei qui ha citato, (con progetti europei, internazionali e nazionali) va bene sempre. Purtroppo, però, si dà il caso che in questa risposta non ci sia niente di concreto, cosa che è grave da questo punto di vista: noi possiamo discutere dell'acqua su Marte, basta non farlo in relazione agli assetati, facendo loro credere che potranno, pazientando solo un po', berla. Stiamo allora alla sete di energia che hanno il nostro Paese e la nostra economia e rinunciamo a portare la discussione sul passato referendario dell'Italia, sulla sicurezza e sulla difficile gestione delle scorie che ancora non risolviamo dal 1987. Stiamo solo ai due più brutali parametri: tempi e costi. la centrale di Olkiluoto in Finlandia ha visto approvato il suo progetto nel 2000 ed è entrata in funzione nel 2022, per due mesi soli, perché a dicembre scorso hanno trovato materiale estraneo nel reattore. Ci sono voluti Noi non siamo nemmeno all'anno zero, visto che qui anche oggi non abbiamo parlato di un progetto, ma solo di ricerche. Il costo per la Finlandia è stato di 8,5 In teoria, questa centrale dovrebbe produrre 13 TWh l'anno, lo stesso di 10 gigawatt di fotovoltaico, che alla media dell'attuale produzione italiana richiederebbero tre anni, in crescita progressiva ovviamente. Perché la centrale nucleare produce zero energia finché non è del tutto realizzata. Il costo di 10 gigawatt di fotovoltaico è di 6,5 miliardi, più i sistemi di accumulo. Di capitali privati però. Lo ha spiegato bene di recente l'associazione Elettricità Futura, anche alla presenza, oltre che del ministro Urso, del ministro Pichetto Fratin. Mentre i privati nel mondo e in Europa sono ormai usciti dal nucleare, al netto del grande Charles Montgomery Plantageneto Burns, che lei conoscerà. quindi di un investimento pubblico di almeno 8,5 miliardi per un impianto che forse fornirà energia tra ventidue anni. Il senatore Cottarelli ha presentato un ottimo disegno di legge sulla trasparenza dei programmi elettorali, per questo facevo riferimento alla serietà della politica. politica. Il disegno di legge dice che si devono fornire adeguate informazioni quantitative sul costo delle misure proposte e sulle relative coperture. Questa è la serietà della politica: dire nel programma elettorale che si vogliono realizzare centrali nucleari per rispondere alla crisi energetica e dire poi dove si realizzeranno, con quali tempi e con quali costi e non, invece, far passare le elezioni e dichiarare quello che già sapevamo, che esistono progetti di ricerca che richiederanno anni e anni. Se non verrà in nostro soccorso una legge - e concludo - spero che verrà in nostro soccorso una bella massima attribuita a Lincoln: «Si possono ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non si possono ingannare molte persone per molto tempo».

dell'ambiente ha prontamente provveduto ad acquisire informazioni circa quanto descritto nell'interrogazione. Pertanto, il Comune di Fossalta di Piave rappresenta che, con provvedimento del 16 novembre 2018, veniva posto sotto sequestro penale un capannone industriale sito in via delle Industrie, nn. 14-16, con tutto il suo contenuto, in quanto veniva accertato che all'interno di suddetto capannone albergava un deposito abusivo di rifiuti. Di più, a causa dei costi giudicati notevoli per le operazioni di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti, il Comune precisa che non è stato ancora possibile attribuire con precisione i codici d'identificazione degli stessi rifiuti. Purtuttavia, risultano concluse le indagini sul piano giudiziario, nonché individuati i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda; segnatamente, parte di essi ha avuto accesso al rito abbreviato, mentre per altri risulta ancora in corso il processo presso il tribunale di Milano. Come ricordato dall'onorevole interrogante, il Comune di Fossalta ha provveduto a emettere le ordinanze per cui, in caso di inottemperanza, è previsto l'intervento sostitutivo d'ufficio in danno dei soggetti responsabili, ai sensi dell'articolo 192 del testo unico ambientale. In particolare, le ordinanze emesse sono state tre e i relativi termini di adempimento sono scaduti. Se il Comune stesso si è attivato in sostituzione dei soggetti inottemperanti per quanto indicato in due delle tre ordinanze, per quanto riguarda l'ultima concernente la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti - l'ente rappresenta di non essere nella condizione di agire analogamente a causa dei costi stimati per le operazioni previste che eccedono assolutamente la disponibilità e la capacità di spesa del Comune. Pertanto, risulta chiaro che il problema risiede nel reperimento di fondi sufficienti per il corretto ripristino delle condizioni del capannone. A questo proposito, si apprende altresì che, anche attraverso interlocuzioni con le istituzioni locali, al momento le stesse non hanno dato adeguato riscontro alla richiesta di congruo sostegno economico Nel condividere pienamente le preoccupazioni espresse riguardo le potenziali criticità che potrebbero derivare dalla situazione descritta, si sottolinea come il Ministero non abbia la competenza specifica per intervenire nel caso di un deposito abusivo di rifiuti in prossimità di un centro abitato. Tuttavia, attesi un procedimento giudiziario in corso e la prevalente competenza di soggetti quali la Città metropolitana di Venezia, la Regione e la Provincia, il Ministero dell'ambiente si rende disponibile a valutare l'opportunità di partecipare a un incontro che possa essere funzionale alla sensibilizzazione di tutti i soggetti preposti nell'identificare lo strumento più idoneo per il ristoro del Comune di Fossalta di Piave.

da lei rappresentato si è messo tempestivamente in azione per verificare cosa sia possibile fare per risolvere questa difficile situazione, che appare come un fatto specifico, ma in realtà ha una dimensione davvero particolare, che merita l'attenzione anche del Ministero dell'ambiente, nonostante lei abbia detto che il Dicastero che rappresenta non ha le competenze esclusive per risolvere la questione. Fossalta di Piave è un bellissimo Comune, sul fiume Piave, della città metropolitana di Venezia e si è trovato a vivere questa situazione proprio perché nelle vicinanze del centro c'è un capannone nel quale sono state stoccate circa 10.000 balle di rifiuti non identificati. Ciò desta una preoccupazione legittima nelle istituzioni locali e nei

Parlamento, come Governo e istituzioni locali, di reperire le risorse affinché il Comune possa intervenire e procedere con un'azione di bonifica. Se poi dovesse ritenere, signor Sottosegretario, che nell'ambito dei suoi impegni istituzionali sia possibile anche

e penso di poter parlare anche a nome delle istituzioni locali - nella leale collaborazione sua e del Governo per fare in modo che si possa risolvere il problema, rassicurando tutta la comunità di Fossalta di Piave.

cui risultano sottoposte persone e cose in caso di eventi alluvionali, chiedendo altresì l'opportunità di ripristinare la struttura di missione ItaliaSicura per il contrasto al dissesto idrogeologico. A tal proposito risulta che, con il decreto n. 501 del 22 novembre 2017, dell'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica venne approvato l'elenco degli interventi ricadenti nella Regione Liguria, la cui progettazione, fino al livello esecutivo, è sostenuta finanziariamente mediante il fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrologico del MASE, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

insieme al Comune di Santa Margherita Ligure, con il quale ha sottoscritto una convenzione di avvalimento nel dicembre 2018. La Regione Liguria rappresenta che nel luglio 2020 è stato approvato il progetto definitivo e sono state avviate le attività propedeutiche alla procedura di gara per l'affidamento del progetto esecutivo, per la quale il commissario si avvale della stazione unica appaltante regionale di Regione Liguria. In relazione alla tipologia di intervento e all'importo stimato per l'opera, nel luglio 2021, si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva attraverso la modellazione *building information modelling* (BIM) o metodologia di modellazione informativa. Successivamente, con due provvedimenti del marzo e del maggio 2022, il commissario di governo ha perfezionato l'approvazione dei documenti tecnici di gara e determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il 26 giugno 2022, infine, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, a seguito dell'uscita sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il bando relativo alla gara di affidamento del servizio di progettazione esecutiva con opzione di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del canale scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato nel Comune di Santa Margherita Ligure. Il progetto prevede la realizzazione di un'opera idraulica in galleria di circa 2.400 metri di lunghezza, che dovrà raccogliere e convogliare una parte sostanziale delle delle portate di piena dei torrenti San Siro e Magistrato, al fine di risolvere il problema derivante dall'insufficiente capacità idraulica dei corsi d'acqua che attraversano il centro storico di Santa Margherita Ligure. Il costo complessivo dell'intervento, così come evidenziato dall'interrogazione, inizialmente stimato in 33 milioni di euro, anche a causa dell'andamento dei prezzi delle materie prime, è stato rideterminato in circa 40 milioni di euro. Si rappresenta che le risorse finanziarie non sono rinvenibili nelle dotazioni PNRR affidate alla gestione del MASE, con particolare riferimento alla misura M2 C4, subinvestimento 2.1 (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) che e delle finanze del 6 agosto 2021 - è destinata solo al finanziamento di progetti in essere, ovvero già inclusi in precedenti programmazioni. Per quanto concerne infine la questione relativa alla *governance* delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, a fronte della riconosciuta necessità di accelerare l'attuazione degli interventi, si evidenzia come nell'ambito del PNRR sia stata prevista una specifica misura M2C4, riforma 2.1, di semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. La riforma, finalizzata a superare le carenze esistenti a livello di *governance* dei rischi idrogeologici evidenziati dalla Corte dei conti italiana, doveva mirare a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase, oltre che a realizzare in via prioritaria interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con il principio del non arrecare un danno significativo e in ultimo rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti. Detta riforma è stata portata a compimento entro il termine fissato dal PNRR, ovvero il 30 giugno 2022, superando favorevolmente il vaglio della Commissione europea. In particolare, la riforma è finalizzata a rafforzare il coordinamento dei diversi livelli di governo coinvolti, razionalizzando i flussi di informazione, oltre a definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione dei progetti, quali le autorità di bacino distrettuali e le strutture commissariali. L'impianto della riforma trova fondamento in un complesso di norme approvato nel corso del 2021 e del 2022, quali i decreti-legge nn. 77 e 80 del 2021 e il DPCM 20 settembre 2021, il decreto-legge n. 152 del 2021 e il decreto-legge la cui messa in discussione precluderebbe l'entrata a pieno regime delle diverse misure sopra descritte e dei loro effetti definitivi, compromettendone l'efficacia, nonché gli impegni che sono stati assunti a livello europeo.

fondamentale per la sicurezza dei cittadini del comune di Santa Margherita Ligure, in grado di risolvere definitivamente il problema dell'eventuale esondazione degli affluenti San Siro e Magistrato, questo Governo non risolverà il problema, perché non sono previsti finanziamenti. Mi stupisce molto che sia venuto a raccontarci cosa sta facendo la Regione Liguria in termini di avanzamento e progettazione, per due ragioni. La prima è che ne ero a conoscenza, quindi la sua sottolineatura è del tutto irrilevante; la è che nelle sue parole non c'è uno straccio d'iniziativa che riguardi il Governo che rappresenta. Penso sia molto grave quello che ha

anche su questo ha chiuso completamente le porte. Ciò che mi preoccupa di più delle sue affermazioni è che ci ha fatto un lungo elenco di decreti del passato per giustificare il fatto che - da ciò che mi pare di capire - non abbiate ancora deciso sull'intento di ripristinare o meno l'unità di missione ItaliaSicura. Perché penso che l'unità di missione ItaliaSicura sia fondamentale? Quest'opera,

dell'ex presidente Conte, di cancellare una delle misure più positive che questo Paese aveva avuto in termini di programmazione sul dissesto idrologico. E sempre voi avete deciso in quest'Aula, con il voto di tutti i parlamentari, che doveva esserci una risposta sul tema dell'unità di missione ItaliaSicura,

anche in Turchia e in Siria dovrebbe indurci ad avere un atteggiamento responsabile, serio, pragmatico e di programmazione, sul tema del rischio sia sismico sia idrogeologico. deve arrivare qui in Aula a dire a una popolazione preoccupata che la Regione sta andando avanti sulla progettazione, ma che il Governo non intende mettere un euro né nei finanziamenti esistenti né in quelli del PNRR, e neppure intende decidere o dire che cosa vuol fare per questo Paese su una tematica così importante come la sicurezza dei cittadini. Delle tante volte in cui mi è capitato di ricevere risposta

dato nessunissimo tipo di segnale su nessuna delle questioni poste. Anzi, glielo dico anche in modo molto chiaro: tale risposta, in maniera pilatesca, lascia il problema al livello delle autorità locali. Penso che sia davvero un gesto molto grave. Non sono affatto soddisfatta. Mi auguro che la prossima settimana sulla questione di ItaliaSicura vi sia un pronunciamento

Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di senatori Segretari. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, invito tre senatori Segretari a procedere allo spoglio

alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

della vicenda di cui parliamo. Firenze è una città che continua ad attrarre turismo, ma a dire la verità l'aeroporto di Firenze non attrae soltanto turismo: il 60 per cento dei passeggeri, infatti, è legato a vicende *business.* La questione è molto semplice: Firenze riesce a attrarre a tutti i livelli aziende internazionali e turismo, riesce a fare l'accordo con Pisa le garantisco che l'accordo tra fiorentini e pisani è complicato da qualche secolo, dai tempi di Dante in poi (non mi riferisco all'attualità politica). La conclusione finale è che Firenze fa tutto quello che deve fare, ma oggi una corrente di pensiero antisviluppista e demagogica vorrebbe bloccare l'espansione dell'aeroporto, pensando che se Pisa va avanti, Firenze

è l'unico modo anche per Pisa di poter andare avanti, perché se Firenze viene messa in difficoltà salta anche Pisa? In secondo luogo ho una

Intendete prorogare le misure del decreto-legge sblocca Italia per il sistema aeroportuale? La terza domanda è un po' più provocatoria, me lo consentirà. Visto che dite sempre di voler cambiare il PNRR

L'aeroporto di Firenze è un aeroporto di rilevanza strategica, come dovrà tornare a essere quello di Pisa e su questo il Ministero sta lavorando e possono, anzi devono, crescere entrambi. Non esiste l'uno che va avanti a discapito dell'altro. Io personalmente, il mio movimento e il Governo, siamo a favore dell'ampliamento, dello sviluppo e della crescita dell'aeroporto di Firenze e del sistema aeroportuale toscano. Ovviamente, nella risposta per lei e per chi ci sta coraggiosamente seguendo da casa, tutto l'*iter,* che vede il *masterplan* che va a conclusione entro il 2023, nonostante ci siano rilievi da parte di alcuni Comuni. Penso al Comune di Prato e penso al Comune di Sesto Fiorentino. Io mi sono proposto come il Ministro dell'ascolto dei sindaci e dei territori, ma son convinto che il contributo del Ministero, della Regione e dei Comuni, con opere compensative, potrà portare a un accompagnamento di tutto il territorio, a una crescita dovuta, doverosa e naturale dell'aeroporto di Firenze come parte integrante del sistema aeroportuale. Stiamo valutando l'utilizzo di tutte le opportune semplificazioni procedurali, compreso lo sblocca Italia, il cui principio è ampiamente ripreso dal nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici, che ho avuto l'onore di portare in Consiglio dei ministri nel nome della modernizzazione e che quest'Aula dovrà approvare entro il 31 marzo. Son convinto che Firenze potrà vivere un grande momento di sviluppo. È stato appaltato oltre un miliardo di lavori per la stazione la tramvia, che ovviamente arriverà a conclusione. Aggiungo una mia riflessione: ciò avverrà senza penalizzare il traffico privato. Quindi, incentivare il trasporto pubblico locale, sì; però, scudi verdi, ZTL estese, penalizzazioni patrimoniali e tasse d'ingresso a Firenze come a Milano non mi convincono e non aiutano il futuro. Sulla rimodulazione del PNRR sfonda una porta spalancata. Abbiamo trovato delle poste di bilancio che non saranno mai esaurite. Il buon senso potrà e dovrà portare a ricontrattare con l'Europa, per andare a girare queste risorse laddove vengono richieste. Il tema aeroporti, dal mio punto di vista, è un tema che assolutamente dovrà e potrà ricadere in questo ribilanciamento dei fondi PNRR. Quindi, può crescere Firenze, può crescere Pisa, può crescere la Toscana, può crescere l'Italia intera. Signor Presidente, io sono molto soddisfatto della risposta del signor Ministro. la città di Firenze attrae aziende, turisti, cuori padani. Quindi, siamo contentissimi di questo. Però, il punto fondamentale che io volevo sottolineare è proprio quello che il Ministro ha detto: se Firenze non cresce, Pisa è finita, anche se su questo credo che non tutti qui siano d'accordo. Apprezzo molto il fatto che abbiate cambiato idea sullo sblocca Italia. Anzi, dopo averlo contestato, sia sulle trivelle che, in questo caso, sugli aeroporti, siete in prima linea per

al singolo Vice Presidente del Consiglio, ma al Governo. Noi siamo sicuri che col ministro Salvini questo problema non si verificherà, ma è accaduto che, con le stesse interrogazioni, con i cosiddetti *question time*, il Governo sia venuto in Aula e ci abbia detto alcune cose. Mi riferisco al ministro Abodi sulla famosa vicenda dei 900 milioni regalati dal Governo alle società di serie A. Il ministro Abodi è venuto qui e ha detto: non vi preoccupate, non ne faremo niente. Poi, invece, avete votato a favore della norma che ha dato 900 milioni alle società di calcio di serie A. Io mi auguro che stavolta gli impegni che avete preso in Parlamento, e che io condivido, li rispettiate. Sarebbe assurdo che, dopo che il Ministro è venuto qui a prendere degli impegni, facesse come ha fatto il ministro Abodi, rimangiandosi la parola per fare un regalo alle società di calcio. Ma sono certo che non accadrà.

dell'itinerario internazionale che va da Civitavecchia fino a Mestre, ma soprattutto è importante per l'economia dei territori della Tuscia, un territorio che abbraccia la ragione Umbria, parte della regione Lazio e che sconta ancora gravi ritardi infrastrutturali. L'area del Viterbese, di grande pregio turistico e con tanti insediamenti produttivi e artigianali, soffre per questa carenza di collegamento, così come tutta l'area nord della Regione Lazio, che avrebbe bisogno di servizi migliori. Le aree interne devono essere dotate di migliori infrastrutture collegate al mare e all'importante porto di Civitavecchia, che peraltro si trova al centro

per l'accesso alle più importanti zone turistiche italiane e alle grandi rotte crocieristiche del Mediterraneo. Diversi tratti di strada sono stati realizzati fino a Monte Romano, ma il mancato completamento dell'ultimo tratto impedisce il pieno utilizzo di quella che è considerata a tutti gli effetti una infrastruttura strategica. Per ultimare il nuovo svincolo di Monte Romano Est risultano già stanziati 355 milioni. Ricordiamo che il completamento di quest'opera

però stiamo correndo. Il collegamento Orte-Civitavecchia è di fondamentale importanza per il Paese, come lei ricordava. Come Ministero abbiamo dato 35 milioni di euro di contributo al Comune di Civitavecchia per l'ampliamento di un porto fondamentale per tutto il Lazio e per il recupero di alcune aree dismesse in città. Quindi il completamento della Orte-Civitavecchia, per quanto ci riguarda, è fondamentale. Senatore, la parte di cui lei parlava, da Monte Romano fino alla costa tirrenica, è costituita dalla strada statale Aurelia bis, che risulta oggi evidentemente inadeguata alla domanda di traffico, perché a carreggiata singola e con una corsia per senso di marcia. Per realizzare l'adeguamento dell'intero collegamento stradale fino al congiungimento con la dorsale tirrenica è stato nominato un commissario straordinario nel lontano 2021. Il progetto di adeguamento del primo stralcio funzionale, con estensione di cinque chilometri prevalentemente in galleria, è stato approvato con ordinanza del commissario il 31 gennaio di quest'anno. Proprio ieri, l'Anas ha pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il bando per l'esecuzione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'intervento, con un valore complessivo dell'appalto di 285 milioni di euro. Relativamente al secondo stralcio, compreso tra Tarquinia e Civitavecchia (innesto con sono in fase di avvio i tavoli di concertazione per il completamento dell'opera. Questo è uno dei 117 interventi commissariati che ho trovato cento giorni fa sulla mia scrivania e che, le posso assicurare, troveranno compimento nei tempi previsti recuperando i vent'anni perduti. La ringrazio per l'interrogazione e spero che lei e chi ci sta seguendo da casa nell'area del Nord Lazio possiate tenere la registrazione di quanto ci siamo detti fino ad oggi, e poi magari andremo insieme a inaugurare la conclusione dell'opera. la ringrazio, sono soddisfatto della sua risposta e, come parlamentare eletto in quei territori, accolgo volentieri l'invito a inaugurare queste opere non appena saranno completate. Del resto, questo tratto è famoso. L'Aurelia è celebre e anche il film «Il sorpasso» è ambientato su quel tratto di strada, con un epilogo che ovviamente fu molto amaro; invece, noi speriamo in un *happy end* di realizzazione di infrastrutture, che sono importanti - lo sottolineo - perché collegano il porto di Civitavecchia che è fondamentale anche per l'attività turistica, crocieristica e non solo italiana; è un collegamento fondamentale verso la Sardegna, quindi garantisce una continuità territoriale attraverso il mare. mare. L'area di Orte e dintorni collega l'Umbria, che è un'altra Regione che per ragioni geografiche trova tante limitazioni, essendo collocata nel cuore dell'Italia, con tante bellezze ma ha la necessità di un accesso anche agli sbocchi al mare. Credo che sia importante quello che lei, Ministro, ci ha riferito, peraltro aggiornato fino a ieri con la pubblicazione dei bandi, quindi diciamo che il *question time* questa volta è *in time* perché l'aggiornamento è rilevato alla giornata di ieri. La ringrazio ancora e mi auguro che quest'opera sia completata, come tante altre, nell'azione che sto seguendo e che apprezzo, insieme a tanti italiani, di concretezza per la politica del fare.

Signor Ministro, la doppia transizione verde-digitale rappresenta la principale sfida per il settore dei trasporti e la competitività europea. Il pacchetto di misure "Fit for 55", adottato dalla Commissione, è finalizzato proprio a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni entro il 2030. Ma, tra gli altri provvedimenti, proprio lo scorso 14 febbraio, il Parlamento europeo ha concluso l'*iter* di adozione del Regolamento CO2 Auto, che prevede l'uscita dal motore endotermico entro il 2035. Sempre nella stessa giornata la Commissione ha poi adottato una proposta di revisione del regolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli pesanti che va nella stessa direzione. Sono infine in fase "trilogo" i tre provvedimenti normativi sull'uso di combustibili alternativi per il trasporto terrestre, marittimo e aereo. Il mercato dell'auto in Italia è essenziale per la crescita del Paese e ha anche dimostrato nel tempo di essere uno straordinario volano dell'economia nei momenti di ripresa dalla crisi. Una transizione verso la mobilità elettrica al ritmo previsto dal "Fit for 55" renderà ovviamente difficile la trasformazione del settore e della sua forza lavoro senza traumi, perché nel solo ambito delle forniture automobilistiche gli obiettivi di CO2 proposti dalla Commissione europea hanno già messo a rischio 500.000 posti di lavoro. Un rischio che si concentrerà maggiormente tra il 2030 e il 2035. Inoltre, l'elettrificazione della mobilità comporta anche il pericolo - di non poco conto - di creare dipendenza dalle importazioni di materie prime e batterie, mantenendo così la creazione di valore al di fuori dell'Unione europea. quindi evidente che la mancanza di una progettualità chiara che consenta alle migliaia di aziende italiane di adeguarsi gradualmente all'imposizione dell'Unione europea rischia di disperdere tutte quelle competenze che si sono fino ad oggi create. create. Ministro, le chiediamo quali iniziative di competenza intenda adottare per rispondere alla sfida della doppia transizione nel settore del trasporto privato e pubblico, anche eventualmente considerando una *road map* mobilità e trasporti,

Presidente, penso che a tutti stia a cuore la qualità dell'aria come dell'acqua e avere un ambiente più pulito, in quest'Aula a prescindere, da destra a sinistra, e a casa. Avere un ambiente e un'aria più puliti, però, non significa licenziare milioni di di operai e far chiudere migliaia di aziende. L'integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio nonché un regalo alla Cina un suicidio dell'Italia e dell'Europa ed è un regalo al gigante cinese. Basta guardare i dati di vendita del 2022; basta farsi delle domande. L'elettrico non è solo la colonnina

senza distruggere un settore industriale e imprenditoriale, anche perché l'elettrico, come dicevo, non è solo la colonnina. Per arrivare alla colonnina, per arrivare alla barriera elettrica devi scavare, inquinare; devi sfruttare in Africa, in Continenti euroasiatici. Quindi, o i sostenitori del "tutto elettrico", che, purtroppo ci sono anche in questo Parlamento, ignorano le conseguenze del tutto elettrico,

per avvantaggiare il gigante cinese mi sembra la follia. Io sto lavorando: ho incontrato il Ministro tedesco, ho incontrato ieri il ministro rumeno ai trasporti, con cui siamo in totale accordo: serve più tempo; servono contributi economici; servono aiuti per chi vorrà cambiare la macchina - che va incentivato e per chi vorrà sistemare casa sua nel nome dell'efficienza energetica. Anche in quel caso, se Bruxelles impone una patrimoniale sulla casa e sull'automobile riuscirà a far inimicare le tematiche ambientali alla maggior parte degli italiani che rischiano di perdere un lavoro. è fondamentale andare avanti sulla via della transizione, senza però, mentre cerchiamo di liberarci dalla dipendenza dalla Russia per il gas, avviarci a una nuova e ben più pericolosa dipendenza dalla Cina per muoverci e lavorare nei prossimi decenni.

il programma di azioni che lei e il Governo metterete in campo di qui a breve, sempre in linea con l'attenzione e la sensibilità che lei dimostra verso i territori e i cittadini. Infatti, giustamente dobbiamo migliorare la qualità del lavoro e della loro vita, promuovendo l'innovazione tecnologica e la sostenibilità, ma nel contempo dobbiamo rafforzare il nostro tessuto imprenditoriale. Sicuramente ciò che le chiediamo, nell'interesse delle e dell'intera società italiana, è che questo tessuto imprenditoriale non venga danneggiato. Il comparto dell'*automotive* è uno dei principali settori strategici del nostro territorio e colpirlo così pesantemente in nome della sostenibilità ambientale significa colpire duramente la nostra intera economia e, di conseguenza, la stessa vita quotidiana delle famiglie, sia per chi rischia di perdere domani il posto di lavoro, sia per tutti gli italiani che potrebbero incorrere in grosse difficoltà, e non solo per l'ipotizzabile contrazione

per un cambio di direzione. Attendiamo anche di avere garanzie sugli aiuti di Stato e i sostegni alle imprese previsti dalla nuova comunicazione della Commissione europea. Da parte nostra, come Gruppo Lega, continueremo certamente a mantenere alta l'attenzione su questo delicato

indubbiamente è stata messa in discussione nel momento in cui due corti d'assise d'appello in Sicilia hanno annullato i procedimenti delle corti di assise territoriali di Palermo e Messina sentenze, accogliendo l'eccezione della nullità del dibattimento a causa dell'avvenuto superamento del limite d'età dei giudici popolari. Si trattava per la corte d'assise di Palermo di fatti di mafia e per la corte d'assise di Messina di un femminicidio, peraltro realizzato mediante contagio da HIV. C'è un terzo processo, sempre a Messina, da parte della corte d'assise che si è concluso con la condanna dell'imputato per un caso altrettanto odioso di femminicidio e anch'esso rischia di essere annullato; è già stato proposto l'appello con l'eccezione del del superamento del limite d'età dei giudici popolari. Signor Ministro, lei è uomo di legge ed è la seconda volta che in poche settimane mi rivolgo a lei in questi termini. Quindi, lei ben sa che la legge n. 287 del 1951, nell'istituire la figura del giudice popolare della corte d'assise, pone un limite d'età per l'assunzione dell'incarico e la composizione del collegio, ma alcuna disposizione nella legge prevede che al raggiungimento di questo limite operi una decadenza dell'incarico. Tra l'altro, mi permetto di osservare che, se così fosse, i giudici si troverebbero nella necessità di verificare continuamente il requisito dell'età. E, poi, quando li dovrebbero sostituire? Un giorno prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età? Il giorno dopo? Quand'è che si invaliderebbe tutto il processo? Eppure, questa interpretazione, che - ahimè - è andata in senso demolitivo del lavoro della corte e non conservativo, come invece il diritto avrebbe imposto e richiesto, ha travolto già due processi e tanti altri sono a rischio di essere travolti. Allora, la certezza del diritto è questa, signor Ministro: è la certezza dei cittadini che, quando fanno ricorso alla giustizia, quando affidano alla giustizia le loro vicende, tra l'altro dolorosissime, perché i processi di corte d'assise vertono sui casi più importanti di reati verso la persona, non possono poi essere abbandonate all'idea che la giustizia sia come un lancio di dati, oppure sia affidata a interpretazioni che possono cambiare nel tempo e portano alla demolizione di processi importanti,

intende lei promuovere un'indagine in merito ai fatti che le ho illustrato, anche conoscitiva, volta ad accertare quanti processi in corte d'assise si trovino o si troverebbero, se si confermasse questa interpretazione, a rischio di essere annullati? Vorrei sapere inoltre se non intende, considerando che il dettato normativo è chiaro,

È vero che quelle sentenze sono state annullate dalle corti di appello per nullità assoluta, perché la composizione del collegio era in contrasto con la legge. Lei ha riassunto bene i termini del problema e, quindi, non li voglio adesso ripetere. Si tratta di giudici popolari che avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel momento in cui sono stati chiamati a decidere. Quindi, la corte ha ritenuto di annullare per difetto assoluto quelle condanne. Questo è un orientamento consolidato da parte della Corte di cassazione. Avrei qui tutta una serie di sentenze; l'ultima è Cassazione del 6 ottobre 2003. Ce ne sono molte altre, ma le do per lette. Mi creda: è un orientamento costante della Corte di cassazione quello di ritenere che la piena assimilazione della figura del giudice popolare con quella del giudice togato riguardi anche l'età. Così come il giudice togato cessa a tutti gli effetti di essere tale a settant'anni, compreso il sottoscritto, che a suo tempo è stato "rottamato" (come si dice), tanto vale anche per i giudici popolari. L'orientamento consolidato della Cassazione impedisce qualsiasi attività ispettiva, perché le corti si sono adeguate a tale orientamento consolidato e, quindi, a una sorta di interpretazione autentica che danno le sezioni unite della Corte di cassazione. Non bisogna, però eludere il problema; il problema rimane. rimane. Qui si tratta di intervenire in due modi. Il primo è dare un'interpretazione autentica della legge, come lei pare suggerire. Ma io sarei più propenso a una rimodulazione totale della legge: è una legge del 1951 - per chi non lo sapesse

come il sottoscritto; quindi è abbastanza irrazionale che a sessantacinque anni uno non possa esercitare la funzione di giudice popolare. Le posso assicurare pertanto che saranno nostro compito e nostro intendimento non tanto dare un'interpretazione autentica, che potrebbe a questo punto anche complicare complicare le cose, quanto rimodulare completamente la legge, in modo da allineare l'età dei giudici popolari con quella dei giudici togati.

un intervento normativo che uniformi l'età degli stessi. Con riferimento alla vicenda concreta, però, prendo atto delle sentenze della Suprema corte che lei ha citato, ma non mi risulta che ci sia una sentenza a sezioni unite della Cassazione. La procura generale di Palermo ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte d'assise d'appello, proprio perché ha voluto salvaguardare o comunque mettere in discussione tale interpretazione, ritenendola errata. Su questo punto non mi posso dire soddisfatta, perché ritengo che ci possa essere margine per un'interpretazione più aderente - a mio avviso - al testo normativo. La ringrazio invece per l'impegno assunto con la sua dichiarazione.

da un articolo pubblicato sul quotidiano «Domani», nonché su altri organi di stampa, il 14 febbraio del 2023, si apprende che fino al giorno 23 dicembre 2022 i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*, che avevano possibilità di comunicare con il detenuto Cospito, sottoposto al medesimo regime, erano considerati di scarso spessore criminale o, comunque, non costituenti un pericolo attuale. Successivamente questo gruppo di socialità nel quale era inserito Alfredo Cospito è stato modificato. I precedenti detenuti, appartenenti a quel gruppo, sono stati sostituiti da tre *boss* considerati di alto livello nella gerarchia criminale e tuttora pericolosi. Sappiamo che le frasi estrapolate dai colloqui e riportate nella relazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i cui contenuti - come tutti sanno - sono stati letti il 31 gennaio 2023 in Aula, alla Camera, dal deputato Donzelli, si riferiscono esclusivamente a quest'ultimo gruppo di socialità. Di conseguenza si desume che i contatti e i rapporti più intensi tra il detenuto Cospito e i *boss* mafiosi avvengano solo con il cambio del gruppo di socialità e, quindi, dopo il 23 dicembre 2022. Credo dunque, signor Ministro, che sia legittimo domandarsi chi abbia deciso, susseguirsi degli avvenimenti, la sostituzione dei componenti del gruppo di socialità in cui si trovava Cospito e per quali motivi, dal momento che - a mio avviso - appare singolare la coincidenza temporale tra il suddetto cambio, l'inizio degli ascolti e delle trascrizioni delle conversazioni e la loro successiva "rivelazione" - la definiamo così - nell'Aula della Camera dei deputati. Chiedo quindi di sapere se non si intenda acquisire dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ogni elemento utile a chiarire chi abbia deciso di inserire il detenuto Cospito in un nuovo gruppo di socialità, diverso dal precedente, e per quali motivi si sia deciso di affiancare a Cospito tre *boss* della criminalità organizzata considerati attivi e attualmente pericolosi, in sostituzione dei precedenti, che sembrerebbe invece non costituissero più un pericolo particolarmente grave e attuale. PRESIDENTE.

sulla limitata frequenza dei colloqui con i familiari, sui pacchi che arrivano dall'esterno, sulla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti, e così via. Per quanto riguarda Cospito, partiamo da un principio di ordine generale. Sulla scorta del disposto di cui alla lettera *f)* del comma 2-*quater*, dell'articolo 41-*bis* - diamo anch'esso per noto - i detenuti, tutti appartenenti ad associazioni mafiose eversive ovvero terroristiche, sono suddivisi in gruppi di socialità, formati da un minimo di due o tre - secondo le raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - fino a un massimo di quattro; sono ristretti nell'ambito in modo che possono comunicare tra loro e svolgere le consentite attività socio-ricreative nei limiti previsti dall'ordinamento. Tali gruppi di socialità sono formati in base a quanto previsto dalle disposizioni dipartimentali vigenti, a cura del direttore dell'istituto penitenziario. Ogni detenuto, poi, deve poter accedere all'attività trattamentale, che è fondamentale per il necessario tentativo di risocializzazione richiesto dall'articolo 27 della Costituzione. Il poter passare del tempo in socialità non è altro che un'attività trattamentale - ripeto - che è comprimibile negli stretti e indispensabili limiti di cui abbiamo detto prima, ma non è certamente azzerabile. Nel caso di ristretti per reati di mafia, terrorismo ed eversione e sottoposti al regime del cosiddetto carcere duro, i detenuti inseriti nei relativi gruppi di socialità sono per definizione appartenenti a tale tipologia di criminali, con l'indispensabile accorgimento - questo è importante - di evitare i gruppi composti da appartenenti alla stessa consorteria criminale. E questo è intuitivo. Ciò premesso, Cospito - arriviamo al fatto - all'atto del suo ingresso presso la casa circondariale di Sassari, avvenuto il 20 maggio 2022, è stato inserito nel gruppo di socialità con tre detenuti. Risultano peraltro pienamente rispettate dalla competente direzione del carcere di Sassari le indicazioni stabilite dall'articolo 31 della circolare del 2017, che do per nota, per la formazione del predetto gruppo di socialità. In data 25 giugno 2022, per ragioni inerenti la necessità di riorganizzare le turnazioni delle ore all'aria aperta per i detenuti destinatari di ordinanza della magistratura di sorveglianza, è stato rimodulato il gruppo di socialità, sostituendo due dei precedenti componenti con altri due, tra cui il famoso Francesco Presta. In data 24 dicembre 2022 - quindi recentemente Cospito è stato inserito su proposta del responsabile GOM e conseguente disposizione del direttore del carcere di Sassari in un'ulteriore diverso gruppo di socialità, a causa dell'ingresso in carcere di un detenuto che non poteva essere unito, secondo il 41-*bis,* a detenuti della medesima area criminale. È importante sapere però che questa variazione è stata comunicata alla direzione distrettuale antimafia di Torino, che - come sappiamo - è competente *in parte qua* - come ho già riferito a suo tempo sia alla Camera dei deputati e alla direzione nazionale antimafia, con la nota del 30 dicembre 2022. Infine è mio dovere rappresentare come costante e assolutamente attenta sia la vigilanza amministrativa che gli operatori del GOM, che gli operatori del GOM, addetti alla vigilanza e all'osservazione di detenuti sottoposti al regime speciale, pongono in essere anche sui colloqui che intercorrono tra detenuti sottoposti allo speciale regime. Aggiungo che la questione in questo momento è sospesa, per la ragione che tutti sappiamo, ovvero che Cospito è ricoverato in ospedale per tutelarne la ribadisco ancora una volta che, essendo la salute bene primario e irrinunciabile per tutte le persone, è ricoverato in un'area di eccellenza dell'ospedale di Milano, che monitorizza minuto per minuto le sue condizioni di salute.

Devo dire che non mi ritengo minimamente soddisfatto dell'intera gestione della vicenda Cospito, ma lei questo lo sa, perché ho avuto modo di dirlo anche in quest'Aula durante l'informativa che si è tenuta qualche settimana fa. settimana fa. Non sono però nemmeno soddisfatto della risposta specifica che lei ora mi ha dato. Ovviamente conosco la circolare del 2017, nella quale peraltro si dice, in maniera molto precisa, che andrebbero evitati contatti tra personaggi di spicco, preferendosi che i gruppi siano formati da un personaggio di spessore e altri di minor calibro. Credo che alla domanda che le ho rivolto la sua risposta non sia soddisfacente, perché non ho ancora capito le ragioni del cambio di gruppo di socialità il motivo per cui a un certo punto il gruppo è stato composto da quattro persone, ovvero da Cospito con tre *boss* considerati oggi di altissima pericolosità criminale. Devo dirle che continuo a considerare molto singolare, o perlomeno curiosa, questa coincidenza - chiamiamola così - e cioè l'assenza di comunicazioni nei due mesi precedenti il fatto che Cospito abbia cambiato gruppo di socialità, nonostante fosse in sciopero della fame già da due mesi, e quindi nonostante ci trovassimo dinanzi a una situazione perlomeno eccezionale Insomma, mi pare di poter dire che, nella migliore delle ipotesi, questa sia stata perlomeno una grave

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, da fonti di stampa si apprende che la Corte di cassazione ha anticipato al 24 febbraio l'udienza in cui si pronuncerà sul ricorso presentato dalla difesa del detenuto Alfredo Cospito contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva confermato il regime di cosiddetto carcere duro, ai sensi dell'articolo 41-*bis*. Sempre da fonti di stampa si apprende che gli uffici giudiziari chiamati a esprimere un parere sulla revoca del 41-*bis* ad Alfredo Cospito sarebbero divisi. divisi. Per esempio, l'ANSA il 2 febbraio scrive, che mentre la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo apre uno spiraglio sulla possibilità di far tornare l'anarchico al regime dell'alta sicurezza, sia pure con tutte le cautele del caso, la procura generale di Torino non vede altra strada che la forma del carcere duro. Pure in presenza di valutazioni apparentemente discordanti, il Ministro interrogato ha deciso il 12 gennaio di rigettare la richiesta di revoca del regime di carcere duro avanzata dalla difesa di Cospito. Sul quotidiano «la Repubblica» del 13 febbraio 2023 si legge la procura generale della Cassazione non la pensa affatto così e chiede al tribunale di sorveglianza di Roma di rivedere la decisione sul 41-*bis.* Attenzione alle date, signor Ministro: il 9 febbraio Nordio ufficializza il suo sì al carcere duro. Peccato che il giorno prima il sostituto procuratore della Corte, Piero Gaeta, depositi l'atto che libera Cospito dal 41-*bis.* Sempre nell'articolo viene raccontato che: «L'unico a non aver letto il parere del procuratore generale della Cassazione su Alfredo Cospito, che di fatto lo libera dal 41-*bis,* è Carlo Nordio. Lo leggerà solo oggi se lo riceverà nel suo ufficio di via Arenula». Il presente interrogante chiede quali siano le ragioni che hanno determinato il Ministro al mantenimento del regime differenziato per Alfredo Cospito e se la requisitoria del procuratore generale della Corte di cassazione sia pervenuta ai suoi uffici.

come ho detto anche alla Camera e precedentemente in Senato, il regime cui è sottoposto Cospito poggia su due procedimenti: primo è di esclusiva competenza giurisdizionale e pende attualmente presso la Corte di cassazione, salvo un rinvio alla Corte costituzionale; l'altro poggia su una richiesta di revoca dell'articolo 41-*bis* avanzata dal difensore di Cospito direttamente al Ministero. Per quanto riguarda questa seconda richiesta, i presupposti per la revoca sono quelli della sopravvenienza di fatti nuovi e la sopravvenienza di fatti nuovi fatti nuovi che legittimassero la modifica è stata esclusa radicalmente

prospetta l'eventualità di un trattamento diverso per Cospito. Ma, per quanto riguarda le ragioni di diritto che avrebbero legittimato alla revoca, il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è nettissimo: sono assolutamente fallaci. Questo per quanto riguarda quel 41-*bis* che concerne l'attività ministeriale. La seconda parte, o meglio la prima parte, che riguarda l'attività giurisdizionale, contemplava e contempla un parere della procura generale della Corte di cassazione rivolto alla Corte di cassazione. Questa è esclusiva competenza della magistratura autonoma e indipendente, sulla quale il Ministero non può e non deve avere alcuna interferenza. Il parere della procura generale della Corte di cassazione non poteva e non doveva essere inviato al Ministero, perché è un atto endoprocessuale. Questo Ministero ovviamente non era a conoscenza e non poteva esserne a conoscenza; se ne fosse stato a conoscenza, sarebbe stata evidentemente una violazione della procedura ordinaria; ne è venuto a conoscenza attraverso la stampa, come spesso accade. Pertanto quell'articolo del quotidiano «la Repubblica» è completamente infondato, perché il Ministero non era a conoscenza del parere della procura generale della Cassazione, e non poteva e non doveva esserne a conoscenza. il parere della procura generale della Corte di cassazione non è stato, non poteva e non doveva essere inviato al Ministero che si occupa di tutt'altra cosa. Che poi sia uscito sulla stampa, con quelle rappresentazioni che non esito a definire fasulle, è un'altra questione. Come spesso accade, anche noi veniamo a conoscenza dalla stampa di atti che dovrebbero essere riservati.

Occorre rilevare che proprio una esasperazione del tema, unita a una certa stampa avvelenata, per esempio quella che accusa il Presidente del Consiglio di voler vedere morire in carcere il detenuto Alfredo Cospito, non aiuta il momento che vive il Paese e non aiuta le istituzioni a tutti i livelli. Noi siamo convinti che sul 41-*bis* non si arretrerà di un centimetro. Lo riteniamo un baluardo per la lotta alla mafia. Lo dico da siciliano che ancora ricorda le colonne di fumo che si innalzarono dalla città di Palermo. E ricordo ancora il motto di quella generazione del 1992: contro la mafia lotta con noi. Era un vecchio un vecchio *slogan* del Fronte della gioventù. Quindi, sono convinto che su questa battaglia non torneremo indietro. Non mi resta che ringraziarla per il suo intervento e dichiararmi assolutamente soddisfatto.

onorevoli colleghi, oggi pomeriggio pongo all'attenzione dell'Aula e del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un tema che ritengo sia di interesse per molti cittadini che ci stanno sicuramente seguendo da casa. Mi riferisco al reddito di cittadinanza. Secondo i dati ufficiali del 2022, sono stati spesi quasi otto miliardi per finanziare questo strumento. Da quando è stato introdotto, invece, sono stati spesi complessivamente oltre 25 miliardi di euro. Nel corso del tempo, inoltre, abbiamo visto emergere, purtroppo, con costanza i casi dei cosiddetti furbetti. La cronaca, infatti, ci porta quotidianamente a persone che beneficiano di questa misura assistenziale senza averne il diritto. Penso ad esempio alla recente operazione dell'Arma dei carabinieri, che ha portato alla scoperta di una truffa ai danni dello stato pari a 430.000 euro da parte di alcuni esponenti dei *clan* Casamonica e Spada. e Spada. Ancora poche settimane fa, a Catanzaro la Guardia di finanza ha scoperto 150 persone che illecitamente percepivano il reddito. La misura, così come è stata concepita, rischia di trasformarsi in un vero e proprio freno al lavoro e, infine, si presta alle più disparate forme di raggiri ai danni delle casse dello Stato. A dimostrare oggi il fallimento sono anche e soprattutto altre cifre. I numeri, purtroppo, parlano da soli. Tra i beneficiari del reddito, infatti, ben 404.000 sono considerati occupabili. Dall'altro lato, le aziende oggi cercano 500.000 lavoratori secondo un rapporto di Anpal e Unioncamere. saremmo a pari tra quelli che sono occupabili e il lavoro che viene cercato dalle aziende. Secondo un ulteriore studio, più della metà dei percettori del reddito di cittadinanza che avevano ricevuto un'offerta di lavoro aveva deciso di non accettarla, mentre addirittura il 53 per cento motivava il rifiuto dell'offerta perché non in linea con le proprie competenze. Sono tutte persone che potevano andare a lavorare e invece continuano a ricevere il sussidio. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza, i recenti interventi in manovra hanno ridotto gli effetti distorsivi di questa misura. Come sappiamo, infatti, il sussidio non andrà più a chi si rifiuta di lavorare. Chiaramente, però, l'attenzione va soprattutto a salvaguardare chi vive in situazioni di disagio, come più volte ha ricordato lei, signor Ministro. Come vi dicevo prima, le aziende richiedono 500.000 lavoratori che sono introvabili. La vera sfida, dunque, è dare non il sussidio, ma il lavoro. il lavoro. Il lavoro è e resta per noi l'unica porta d'ingresso che può portare ciascun cittadino a costruire il proprio futuro, la propria casa, i propri progetti. Al signor Ministro in Aula chiedo come il Governo come il Governo intenda agire per risolvere definitivamente tali distorsioni e quali iniziative intenda avviare per rendere maggiormente efficaci i controlli ed evitare, dunque, che il sussidio sia dato a chi non ne ha diritto.

sociali*. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante perché mi consente di trattare uno degli aspetti più controversi del reddito di cittadinanza, che io ho deciso di affrontare come priorità sin dal giorno del mio insediamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ogni sussidio - come è stato correttamente ricordato - può essere erogato dallo Stato solo grazie alla disponibilità di cassa che si forma con il flusso di imposte. È compito delle istituzioni vigilare affinché nessun sussidio sia erogato a chi non ne ha effettivamente diritto e intervenire per sanzionare in modo deciso chi, frodando lo Stato, di fatto sottrae risorse in particolare ai soggetti più bisognosi di sostegno. A questo proposito, consentitemi di rivolgere un sentito ringraziamento al personale ispettivo, alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine che quotidianamente operano per fare in modo che anche in questo ambito emerga ogni azione illegale e fraudolenta, e non sono affatto poche. Quelli che vengono definiti troppo generosamente furbetti, in verità, hanno avuto ampi spazi di manovra per incunearsi nel sistema di controlli sull'erogazione del reddito di cittadinanza. Per me è emersa sin da subito l'urgenza di iniziative incisive e tra queste segnalo che lo scorso 13 febbraio si è riunita, su mia convocazione e da me presieduta, la commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza presso il Ministero, un organismo strategico che vede la presenza di tutte le autorità ispettive, delle parti sociali e degli enti vigilati. era fermo dal 2018 e non è intervenuto sulle nuove esigenze sorte a seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza. Stiamo rafforzando la capacità di programmazione delle attività di controllo, puntando a obiettivi annuali e prevedendo una maggiore collaborazione con le realtà territoriali e le parti sociali, incrementando la possibilità di sottoscrizione di ulteriori convenzioni e conferenze di servizi tra amministrazioni ed enti per verificare la legittima fruizione della della prestazione assistenziale. Per scongiurare le attestazioni dei nuclei familiari non conformi, con la legge di bilancio 2023 si è intervenuti sulla dichiarazione sostitutiva unica e sono in fase di implementazione, in collaborazione con l'INPS, apposite procedure atte a garantire un migliore utilizzo della precompilazione della dichiarazione, anche mediante la possibilità di interrogare l'anagrafe nazionale della popolazione residente ed effettuare controlli puntuali su altre importanti informazioni. Grazie al potenziamento dei controlli, dunque, solo nel mese di gennaio 2023 sono state respinte 46.250 domande, revocate 7.986 prestazioni e poste in decadenza 14.769 pratiche. In questo senso, anche il documento di programmazione dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2023 prevede un piano di verifiche e contrasto delle irregolarità e delle frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito, tra cui il reddito di cittadinanza. Per sostenere la programmazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rafforza l'efficacia e la capacità operativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso l'immissione in servizio nel 2023 di 1.000 nuovi ispettori, il consolidamento della collaborazione con l'INPS, il Comando dei carabinieri e la Guardia di finanza per le materie di sua competenza. In questo caso è importante il tema della condivisione delle informazioni e il nostro indirizzo prioritario è valorizzare il patrimonio di dati che la pubblica amministrazione può mettere a disposizione. Concludo anticipando che, nell'ambito dei lavori relativi a un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, particolare attenzione è riservata alla gestione e implementazione di ancora più efficaci meccanismi di controllo. intervenire in replica il senatore De Poli,

nella sua formulazione originaria, sulle regole di calcolo del sistema contributivo, ed era erogato a domanda - dico era perché probabilmente adesso è stato profondamente modificato - in favore delle lavoratrici dipendenti autonome che hanno maturato requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021. presupposto per tale anticipo pensionistico era la maturazione dei requisiti di trentacinque anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata, di cinquantotto anni di età per le lavoratrici dipendenti e cinquantanove per le autonome. Considerato che, però, l'articolo 1, comma 292, della legge di bilancio 2023 è intervenuto modificando Opzione donna e riservando a tale misura

estremamente ridotta. Inoltre, solamente alcune donne possono accedere a questo beneficio, ovvero solo coloro che hanno un parente convivente con *handicap* da almeno sei mesi oppure abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento, siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Considerato altresì che la norma, così come inserita, appare discriminatoria - lo sottolineo avuto riguardo alla riduzione delle annualità, laddove la donna sia madre, e i requisiti indicati dalla norma di fatto tagliano fuori un'enorme porzione di platea, in sostanza la percentuale di donne che avevano diritto a questa pensione si è ridotta in modo esponenziale. A fronte delle 20.000 donne - come già detto - che avrebbero potuto usufruire della misura così come originariamente concepita, oggi i numeri di cui parliamo sono ben altri. ben altri. Secondo le stime dell'osservatorio di previdenza della CGIL-Fondazione Di Vittorio, l'attuale platea non corrisponde alle 2.900 donne dichiarate dal Governo in più circostanze, bensì a solo 870 donne. Inoltre, ci sono difficoltà pratiche di applicazione della norma. Le chiedo pertanto di intervenire e come intenda porre rimedio alle difficoltà applicative della norma attualmente vigente, e se intenda adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a eliminare i requisiti restrittivi di accesso alle misure e riportare l'età anagrafica a cinquantotto anni per le attuali lavoratrici dipendenti e a cinquantanove per le autonome, senza alcuna ulteriore limitazione restrittiva per la platea. poi, se intenda chiarire quale sia l'impatto economico effettivo della norma attuale rispetto alla formulazione originariamente prevista, posto che, da studi effettuati, emerge che con la misura di Opzione donna a regime la platea diminuisce con il trascorrere degli anni.

la tematica che coinvolge le lavoratrici donne e la possibilità di conseguire la pensione anticipata. Sull'istituto noto come Opzione donna il dibattito politico e parlamentare è stato nei tempi recenti particolarmente complesso. Opzione donna - come è stato ricordato - è stata introdotta come misura sperimentale già nel 2004: consentiva l'accesso anticipato al sistema pensionistico con requisiti pari a trentacinque anni di contributi e un'età di almeno cinquantasette anni, ed è stata, con il tempo, oggetto di modifiche che hanno visto l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi. Con riferimento all'impatto economico della norma attualmente in vigore, l'articolo 1, comma 292, della legge n. 197 del 2022 - come ricordato - precisa che la platea delle beneficiarie è composta da 2.900 lavoratrici che maturano i requisiti pensionistici nel 2023. Questa platea si incrementa a 4.500 per il 2024 e a 5.100 per il 2025. Questi dati risultano nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma, che dimostra anche come gli oneri della misura

anche in un contesto più organico, nell'ambito di un progetto di riforma delle pensioni, per la cui elaborazione ho convocato un apposito tavolo di confronto con le parti sociali, che si è già riunito il 19 gennaio e il 13 febbraio scorsi. Uno degli obiettivi del mio Ministero e del Governo è infatti evitare il rischio di dover nuovamente intervenire con provvedimenti di breve periodo inseriti nella legge di bilancio. Inoltre, rappresento che proprio in questi giorni ho incontrato alcune rappresentanti del movimento Opzione donna, con le quali abbiamo discusso delle modalità per assicurare alle donne l'accesso pensionistico anticipato, tenendo conto di una carriera che troppo spesso non può essere parificata, anche in termini di durata e di continuità, a quella degli uomini. Concludo assicurando la piena condivisione e consapevolezza della necessità di ampliare la platea delle destinatarie dell'attuale anticipo pensionistico, che deve trovare le adeguate coperture finanziarie. A tal proposito, sono in corso le opportune verifiche degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'intervento attuato con la legge di bilancio 2023, assicuro che stiamo tenendo conto delle segnalazioni relative alle difficoltà applicative della misura e che sono in fase di elaborazione specifiche proposte normative, sottoposte al MEF per la verifica della copertura finanziaria, per la quale confermo la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a concorrere utilizzando risorse del proprio bilancio al fine di una rapida definizione delle misure.

Credo che uno dei compiti di un Governo, nel momento in cui si presenta a governare l'intera Italia, sia quello di non rispondere solamente al suo elettorato,

nella loro vecchiaia e adesso voi, Governo, state togliendo loro questa serenità. La sua risposta, Ministro, è incompleta, perché non ha tenuto conto che gli ordini del giorno del 2018, firmati da Giorgia Meloni, indicavano in Opzione donna una misura da sostenere e da incrementare. Abbiamo degli ordini del giorno: ordini del giorno: quindi il Governo che lei qui rappresenta ha realmente omesso di rappresentare 20.000 donne, che chiedevano nient'altro che dignità nella prosecuzione del loro rapporto pensionistico.

hanno difficoltà a ricevere l'assegno pensionistico. Quindi, non si sono attivati neanche con circolari INPS per definire effettivamente in che modo debbano ricevere questo trattamento pensionistico. Io la sprono però a prendere veramente

Capisco che il tema è ripetitivo, ma è talmente ricco che può offrire molti spunti. Parto dal fatto che noi sappiamo tutti che Opzione donna, per come è stata costruita, è una norma in realtà penalizzante per le lavoratrici. È l'unica forma previdenziale che richiede forme di ricalcolo che riducono la pensione che per gli uomini, ad esempio, non sono state mai individuate. Soprattutto, è penalizzante perché non tiene conto del fatto che le lavoratrici hanno un doppio lavoro, come noto da tempo: quello di cura e quello che si fa nel mercato del lavoro; spesso il primo viene ricondotto alla sola maternità, ma non è solo la maternità. Le donne hanno carriere discontinue e sono quelle che hanno subito il maggior innalzamento dell'età pensionabile attraverso le varie riforme. Allora il primo tema è che le norme che avete introdotto rispetto ad Opzione donna non solo riducono la platea, ma introducono dei criteri discriminatori che poi hanno degli effetti: per esempio, il numero di figli non può determinare un cambiamento del contributo previdenziale; i termini di raggiungimento della pensione devono essere raggiungibili per ognuno non sulla base delle proprie abitudini di vita o delle proprie difficoltà. Lo stesso avete fatto rispetto ai licenziamenti, perché si introduce la differenza tra una lavoratrice che viene licenziata nell'ambito di un tavolo di crisi e una lavoratrice licenziata che non ha accesso a un tavolo di crisi, perché magari è un'azienda più piccola o un territorio meno Da questo punto di vista c'è un primo problema: i criteri discriminatori. Lei, Ministra, si era impegnata il 19 gennaio, nell'ambito del tavolo con le organizzazioni sindacali, a intervenire. È passato il milleproroghe e questo intervento non lo si è visto. Vorrei ricordare che nel frattempo siamo a febbraio e quindi la possibilità delle lavoratrici di decidere cosa fare del loro avvenire è molto seria.

aver proposto il quesito, che ha delle analogie con il precedente, ma che intende evidenziare e chiedere quali interventi questo Governo intende adottare in favore delle donne interessate da Opzione donna. È un tema particolarmente importante e sono consapevole che le donne spesso scontano il peso di carriere lavorative condizionate anche dal lavoro di accudimento e di cura familiare. Come ho già detto in risposta alla precedente interrogazione, l'ultima legge di bilancio ha novellato l'istituto, modificando i requisiti anagrafici e introducendo delle condizioni legate a particolari *status* di bisogno. Ribadisco nuovamente il mio impegno a introdurre nuove forme di flessibilità in uscita a favore delle lavoratrici, nell'ambito di un progetto generale di riordino del sistema pensionistico, che - come ricordava la senatrice interrogante - ha visto la partenza del tavolo lo scorso 19 gennaio, con la convocazione delle parti sociali. Il mio intento è introdurre dei correttivi strutturali per tutelare le carriere contributive di donne e madri, senza dover intervenire annualmente con la legge di bilancio. Al fine di rendere più spediti ed efficaci i lavori di modifica dell'istituto, ho ritenuto importante includere nel confronto anche le rappresentanti del movimento Opzione donna, come dicevo prima. Comunque noi ascolteremo in questo percorso tutti coloro i quali saranno portatori portatori di idee e anche ovviamente di interessi legittimi. Al centro del confronto, oltre alle possibili modifiche del regime di proroga di Opzione donna, c'è anche una riflessione più generale sul tema delle dinamiche di ingresso nel mercato del lavoro e quindi della maturazione dei requisiti pensionistici da parte delle donne. Ribadisco quanto ho già affermato in risposta alla precedente interrogazione in ordine alla necessità che siano individuate, dal Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse necessarie per intervenire sulle modifiche alla misura adottate con la manovra di bilancio e sulla circostanza che questa verifica è attualmente in corso. Voglio quindi rassicurare proposito della mia sensibilità e di quella del Governo e del mio impegno a dare una risposta certa, non solo temporanea, ma di sistema, il prima possibile. Il mio impegno è convinto, come dicevo prima; è per questo che ho offerto anche la disponibilità a concorrere e a sostenere in parte gli oneri finanziari dell'intervento, con risorse presenti nel bilancio del Ministero del lavoro. I tempi sono sicuramente importanti; io lavoro affinché la soluzione sia approntata nei tempi più brevi possibili e mi impegno affinché tutte le circolari e gli atti interpretativi necessari per l'accesso di quelle persone che si trovano nelle condizioni per poter usufruire già dell'intervento così fatto in manovra finanziaria siano immediatamente disponibili. *(Applausi)*. Grazie, Ministro. Le confesso che non mi sento particolarmente soddisfatta di questa risposta, anche se colgo una sensibilità sicuramente interessante. Lei ha parlato di disponibilità a concorrere con le risorse del Ministero rispetto al tema. Vorrei però dirle che c'è una contraddizione, perché o il Ministero è particolarmente ricco, o trovo complesso che esso partecipi della spesa di una vera e propria riforma previdenziale.

che avrebbero bisogno di una risposta adesso e non tra qualche anno. Inoltre, un'esperienza lunghissima, che credo che il Paese ricordi, quella dei cosiddetti esodati, ci ha insegnato che, quando si fa una riforma previdenziale, bisogna avere